La seduta e` aperta (ore 10,32). Invito il senatore Segretario provvisorio a dare lettura del processo verbale della seduta del 29 aprile.

Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha inviato, in data 30 aprile 2008, la seguente lettera di cui do lettura: «Caro Presidente, mi onoro informarLa che la Camera dei deputati, in data 30 aprile 2008, nella sua prima seduta, mi ha eletto Presidente e che, nella seduta stessa, ha avuto luogo il mio insediamento. Con sincera stima e amicizia. F.to: Gianfranco Fini». A nome mio personale e di tutta l’Assemblea rivolgo al presidente Fini i piu` cordiali auguri di buon lavoro. Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento, gli onorevoli senatori hanno indicato alla Presidenza i Gruppi parlamentari dei quali intendono far parte. In allegato al Resoconto della seduta odierna sarapubblicato l’elenco dei componenti di ciascun Gruppo. I Gruppi parlamentari hanno altresı proceduto alla loro costituzione. Gli Uffici di Presidenza risultano essere cosı` composti: Gruppo Il Popolo della Liberta` Presidente: Gasparri Vice presidente vicario: Quagliariello Gruppo Partito Democratico Presidente: Finocchiaro Vice presidente vicario: Zanda Vice presidente: Latorre Gruppo Lega Nord Padania Presidente: Bricolo Vice presidente: Divina Gruppo Italia dei Valori Presidente: Belisario Gruppo UDC, SVP e Autonomie Presidente: D’Alia Vice presidente vicario: Pinzger Segretario: Fosson Gruppo Misto Presidente: Pistorio

dandone comunicazione alla Presidenza entro le ore 17 di lunedı12 maggio. Ricordo altresı che ai sensi dell’articolo 21, comma 4-bis, del Regolamento, i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione Politiche dell’Unione europea saranno designati successivamente alla composizione delle altre Commissioni.

Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, ciascun senatore scriverasulle proprie schede, rispettivamente, due nomi per l’elezione dei quattro Vice Presidenti; due nomi per l’elezione dei tre senatori Questori; quattro nomi per l’elezione degli otto senatori Segretari. Saranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. Al fine di prevenire ogni possibile equivoco, e a disposizione dei senatori, in Aula, l’elenco dei colleghi che hanno lo stesso cognome, con l’indicazione dei rispettivi nomi personali. I colleghi senatori transiteranno sotto il banco della Presidenza per depositare le proprie schede nelle tre distinte urne a tal fine predisposte. Sono chiamati per primi ad esprimere il proprio voto i senatori a vita. La chiama proseguira` con gli altri colleghi senatori in ordine alfabetico. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento, procedo al sorteggio degli otto componenti della Commissione di scrutinio, addetti allo spoglio delle schede.

Dichiaro aperte le votazioni. Invito il senatore Segretario provvisorio a procedere all’appello. GARAVAGLIA

In attesa dei risultati della votazione, sospendo la seduta.

A nome dell’Assemblea e mio personale, desidero rivolgere ai Vice Presidenti, ai senatori Questori e ai senatori Segretari eletti il piucordiale augurio di buon lavoro, non astenendomi dal sottolineare ed apprezzare la forte presenza femminile nel Consiglio di Presidenza, che non riscontro essersi mai manifestata in passato.

Il Senato sara` convocato a domicilio in relazione ai tempi della costituzione del nuovo Governo. La seduta e` tolta